finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni. Avverto che il senatore Giarrusso ha comunicato alla Presidenza di voler trasformare l'interrogazione

senatori, in relazione all'interrogazione della senatrice Ricchiuti, rappresento che il sopralluogo effettuato lo scorso 9 luglio dal personale della DIGOS presso il lido balneare balneare Playa Punta Canna ha consentito di accertare la presenza di diversi cartelli, tra cui uno con la riproduzione di immagini di Benito Mussolini e altri con frasi del signor dipendente del citato lido, che invitavano gli ospiti all'ordine, alla pulizia e alla disciplina. Ulteriori verifiche effettuate sulla rete Internet hanno permesso di individuare anche un video della spiaggia, che riproduceva la voce dello stesso Scarpa mentre pronunciava frasi contro la democrazia. Al riguardo evidenzio che l'ordinamento giuridico prevede - lo ricordo più a me stesso che a lorsignori - alcuni fondamentali presìdi di legalità per la prevenzione e il contrasto di manifestazioni o comportamenti xenofobi e razzisti e, più in generale, contrari al divieto di riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Faccio riferimento innanzi tutto alla legge n. 645 del 1952, cosiddetta legge Scelba, e al decreto-legge n. 122 del 1993, convertito dalla legge n. 205 del 1993, cosiddetta legge Mancino. Gli istituti delineati da tali normative sono oggetto di rigorosa e puntuale applicazione da parte delle autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle forze di polizia. Ciò è avvenuto anche nel caso oggetto dell'interrogazione; il 10 luglio, infatti, il giorno successivo all'invio degli elementi acquisiti dalle forze di polizia in seguito al citato sopralluogo, il prefetto di Venezia ha adottato l'ordinanza, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con la quale è stata intimata al signor Scarpa l'immediata rimozione di ogni riferimento al fascismo contenuto in cartelli, manifesti e scritte presenti all'interno dello stabilimento, con contestuale ordine di astenersi dall'ulteriore diffusione di messaggi contro la democrazia. Sempre nella stessa giornata, il signor Scarpa è stato sentito quale persona informata sui fatti dalla DIGOS e successivamente deferito in stato di libertà per il reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 645 del 1952. La comunicazione di notizia di reato ha portato all'instaurazione di un procedimento penale e il pubblico ministero titolare del fascicolo ha delegato la DIGOS medesima a effettuare ulteriori approfondimenti investigativi. Il rapporto della questura e l'ordinanza del prefetto di Venezia sono stati trasmessi al sindaco di Chioggia per le valutazioni di competenza del suddetto organo amministrativo in ordine all'eventuale revoca della concessione demaniale del lido Playa Punta Canna, rilasciata alla società Summertime Srl. L'ente locale, nel segnalare che, dopo i fatti di luglio, sono stati eseguiti presso il lido in questione diversi sopralluoghi da parte della polizia locale e del personale degli uffici amministrativi, nel corso dei quali non è stata riscontrata la presenza di alcun comportamento illecito, né di forme propagandistiche antidemocratiche o inneggianti al regime fascista, si è riservato ogni ulteriore provvedimento all'esito del procedimento penale in corso. Per completezza di informazione, aggiungo da ultimo che al riguardo si è appreso che la procura della Repubblica di Venezia, nella giornata di ieri, ha chiesto al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale l'archiviazione del procedimento penale.

Penso che sia un grave errore, una drammatica sottovalutazione. Mi rivolgo alla magistratura veneziana e dico: «Ripensateci!». La storia insegna che drammatiche sottovalutazioni di situazioni purulente e schifose come quelle dello stabilimento di Chioggia hanno portato a tragedie. Sottovalutare il pericolo non sarebbe prerogativa solo dei magistrati veneziani. Persino Alcide De Gasperi e Benedetto Croce nel 1922 votarono la fiducia al primo Governo Mussolini, pensando che i suoi modi ruspanti non fossero che folklore, salvo pentirsene per l'abisso di abiezione, morte e distruzione in cui il fascismo ci portò. Persino Papa Pio XI - il Papa della mia città, Desio - aveva detto che Mussolini era l'uomo della Provvidenza, salvo anch'egli ricredersi verso la fine

anatomico. Questo è successo quest'anno, colleghi, non cinquant'anni fa. Devo anche ricordare che la sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 1970 ha ha ritenuto legittimi e compatibili con la libertà di opinione i reati di apologia e d'istigazione, a patto che le opinioni espresse non siano idonee a cagionare un pericolo concreto per l'ordine pubblico.

e xenofoba è entrata in Parlamento con il 13 per cento. Il giornalista del quotidiano «la Repubblica», Paolo Berizzi, cui va tutta la mia solidarietà, che indaga sui fenomeni di diffusione di tendenze violente e intolleranti e che rispolverano il ciarpame fascista, è attualmente tutelato dal servizio di Polizia, in ragione delle minacce che ha subito. Prendo atto della risposta del Governo, ma esorto il giudice per le indagini preliminari di Venezia a respingere la richiesta di archiviazione. Non intendo interferire - evidentemente - con la giurisdizione, ma richiamare l'attenzione dei nostri concittadini (compresi i magistrati) su una situazione molto pericolosa per le nostre istituzioni democratiche, che tutti siamo chiamati a difendere. Qualche volta, opinabili tecnicismi giuridici non sono una buona lente per giudicare la realtà cruda dei fatti.

Signora Presidente, con riferimento alle conseguenze dell'incidente verificatosi nella raffineria di Sannazaro de' Burgondi in data 1° dicembre 2016, l'ENI ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico che, in seguito a tale evento, l'impianto Est è stato immediatamente fermato e isolato dal resto della raffineria. All'interno dell'impianto non si è verificata alcuna esplosione e l'incendio è stato significativamente ridotto e posto sotto controllo grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza della società. Grazie poi al tempestivo azionamento di tutte le misure di sicurezza e prevenzione, tutti i lavoratori presenti nell'impianto sono stati allontanati. Sono infine stati trasmessi alle autorità competenti tutti i dati relativi al monitoraggio dell'aria. In relazione alle conseguenze dell'incidente verificatosi in data 5 febbraio 2017, il giorno seguente la società ENI ha informato il Ministero dello sviluppo economico dell'assenza di conseguenze pregiudizievoli per la salute delle persone e l'ambiente, in quanto il fluido incendiato era gasolio già desolforato e il fumo era rimasto contenuto all'interno del perimetro dello stabilimento. Ciò è stato successivamente confermato dai valori registrati dalle centraline interne allo stabilimento, che non si sono mostrati anormali. Anche l'ARPA della Lombardia, con nota del 7 febbraio 2017, ha chiarito che, in seguito all'episodio, non sono stati registrati significativi incrementi di agenti inquinanti, con particolare riferimento al biossido di zolfo e ai composti organici Peraltro, neppure nella fase acuta dell'evento le concentrazioni di questi inquinanti hanno mostrato incrementi significativi. Infine, in data 2 ottobre 2017, l'ENI ha fornito un aggiornamento in merito all'attività di ripristino dell'unità HDS2 coinvolta nell'incidente, tornata in funzione nei primi giorni di luglio 2017. La società ha comunicato di aver eseguito interventi di miglioramento e adeguamento della struttura, come l'installazione di nuova strumentazione di campo e l'implementazione di specifici piani di controllo, definiti a valle di un'apposita analisi di rischio condotta secondo la metodologia RBI (*risk based inspection*). È stata inoltre estesa la protezione passiva delle strutture con il riposizionamento di alcune tubazioni su un nuovo *rack* progettato e costruito in una zona perimetrale dell'impianto. Durante l'attività di taglio e ripristino dell'impianto stesso, non sono stati poi riscontrati fenomeni corrosivi. Con riferimento ai controlli ambientali eseguiti da enti esterni, dall'attività svolta dalla commissione istituita dalla Regione Lombardia per svolgere un'ispezione straordinaria nella raffineria non sono emerse novità rispetto a quanto già comunicato

proporzioni consistenti, e il successivo accenno di incidente, che per fortuna ha soltanto destato allarme, in quanto si è trattato di un boato notturno, che non ha provocato le conseguenze del primo.

agli episodi verificatisi in quei due specifici incidenti, per quanto riguarda quell'impianto - che oltretutto, per la sua collocazione, interessa la Regione Lombardia, ma ovviamente ha ricadute significative sulla confinante Regione Piemonte si percepisce da parte delle amministrazioni locali e delle popolazioni una sensazione di vulnerabilità. Ciò si assomma - come ho accennato nell'interrogazione nell'interrogazione - agli incidenti di cui abbiamo parlato oggi e al verificarsi di una serie di furti di benzina dall'oleodotto che diparte dalla raffineria che hanno causato sversamenti molto preoccupanti, poiché si sono avvicinati, attraverso le falde sotterranee, ad alcuni pozzi in una zona molto vocata all'agricoltura e quindi fortemente connotata da presenze irrigue.

non si concentrino in quell'area e in nessuna parte del nostro Paese e in Europa, ma purtroppo sono episodi cui assistiamo frequentemente. Pertanto, signor Sottosegretario, esprimo questa raccomandazione ulteriore ringraziandola per la risposta.

innanzitutto ci tengo a ringraziarla, anche a nome degli altri sessantadue colleghi cofirmatari, per aver accettato il difficile incarico ricevuto dal Ministero dei beni culturali di rispondere ad una interpellanza - a procedura abbreviata - che giaceva in attesa di riscontro da ben Certamente meglio tardi che mai, seppure nel corso di questi lunghi giorni le situazioni riportate nell'atto che esporrò hanno prodotto - evolvendosi anche in peggio - seri danni ai titolari dei diritti che la SIAE tutelerebbe in via esclusiva in forza dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore. Per questo motivo mi perdonerà se nell'esposizione dell'interpellanza aggiungerò nuovi motivi a sostegno delle medesime richieste all'epoca presentate e successivamente ribadite anche con altri atti di sindacato ispettivo. Ci terrei innanzitutto a chiarire un concetto che pare sfuggire costantemente al Governo nella sede redigente delle norme in materia. La disciplina dei soggetti che gestiscono i diritti e dei titolari dei diritti stessi deve essere necessariamente elaborata tenendo in debita considerazione il ruolo degli utilizzatori delle opere tutelate. Sono gli utilizzatori che trasmettono le opere attraverso i canali radiotelevisivi, che organizzano rappresentazioni dal vivo e a versare i compensi alla SIAE per ottenere la licenza d'uso. Ebbene, la normativa di settore ha lasciato gli utilizzatori nell'incertezza, con il risultato che in moltissime occasioni le somme vengono accantonate e non versate per paura di sbagliare. Cosa devono fare gli utilizzatori quando si vedono recapitare una richiesta di pagamento da soggetti diversi dalla SIAE e, parallelamente, una lettera della SIAE che diffida dal pagare? Il regime di monopolio della SIAE che, di fatto, dura da oltre centotrent'anni nel nostro Paese, poteva essere interrotto, aprendo le porte alla liberalizzazione della gestione dei diritti d'autore e delle licenze a esse connesse, recependo correttamente Una lettera dello scorso anno, sottoscritta da oltre trecento firmatari tra aziende, imprenditori, *startupper* e investitori italiani nel campo del digitale, esortò il Governo a liberalizzare il settore dei diritti musicali. E questo Parlamento, a più riprese e con più mezzi a disposizione (dalle proposte emendative agli ordini del giorno, dagli atti di sindacato ispettivo agli interventi in Aula), ha esortato il Governo ad indirizzare la propria azione verso una progressiva liberalizzazione. Al riguardo, ricordo che lo scorso 30 marzo 2016, nel corso di una audizione presso le Commissioni riunite 7a e 14a della Camera, il ministro Franceschini aveva dichiarato dichiarato come nella direttiva non fosse presente alcuna indicazione su come i singoli Stati debbano organizzarsi, ma vengano riportati semplicemente alcuni principi che devono essere rispettati. Una interpretazione certamente autorevole quella del Ministro, se non fosse che lo scorso 5 settembre 2017, a seguito di un incontro con la commissaria per il digitale Gabriel, lo stesso Ministro ha fatto marcia indietro, impegnandosi (anche attraverso una lettera inviata alla Commissione, che non disponiamo in visione) ad inserire nella prossima legge di bilancio un correttivo al decreto di recepimento della direttiva Barnier (decreto arrivato, peraltro, con più di un anno di ritardo, assicurando all'Italia una procedura di infrazione) che consentirà agli organismi di gestione collettiva di operare direttamente. La scelta che è stata fatta, ovvero quella di assicurare la libera scelta del soggetto al quale affidare la gestione dei diritti, fatto salvo il monopolio riconosciuto alla SIAE, ha inevitabilmente prodotto incertezze giuridiche (è un po' come dire che si può mangiare qualsiasi tipi di frutta, ma poi comprare solo mele). Si chiede pertanto al Ministero di chiarire, una volta per tutte, il regime applicabile a tutti gli utilizzatori che si trovino nella condizione di voler trasmettere o rappresentare opere non tutelate dalla SIAE. Dovranno questi versare i compensi ad un ente diverso, in violazione dell'articolo 180 della legge sul diritto d'autore? O dovranno non versare i compensi, in violazione degli articoli 12 e seguenti della stessa legge? Sulla gestione della SIAE, il presidente Sugar, in audizione alla Camera dei deputati lo scorso 19 settembre 2017, ha riportato dei dati che dovrebbero descrivere un'entusiasmante ripresa della SIAE, mentre le lamentele degli associati restano inascoltate. A fronte di un miglioramento del bilancio e di costi di gestione mediamente più bassi delle consorelle europee (sono parole del presidente Sugar), e di norme che assicurerebbero la trasparenza degli organi amministrativi dell'ente, le modalità di gestione dei diritti d'autore e di relativa ripartizione presentano evidenti squilibri a danno degli artisti minori, con l'effetto che il 65 per cento degli artisti registrati alla SIAE, alla fine dell'anno, sostiene di percepire in ripartizione dei diritti meno di quanto versa all'ente per la quota di iscrizione, a vantaggio degli artisti e degli autori legati a *major* di rilievo. Rimane inalterata un'altra situazione di fatto, ovvero quella dei ben 527 dei 1.257 assunti a tempo indeterminato che che vantano legami di famiglia o di conoscenza. A ciò si aggiungano i poco chiari investimenti che la SIAE intraprenderebbe, non si sa bene con quali somme, come quello citato dall'ADUC nei titoli della Lehman Brothers: oltre 40 milioni di euro andati in fumo. Tutte queste richieste sono rimaste inascoltate. Nelle more della risposta del Governo, tuttavia, ben altri sono i segnali allarmanti sulla gestione della Società italiana autori ed editori. L'Autorità antitrust, infatti, ha avviato lo scorso 5 aprile 2017 un'istruttoria nei confronti della SIAE per accertare l'eventuale abuso di posizione dominante verso i nuovi attori entranti nel mercato e verso i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei diritti d'autore. Nel provvedimento dell'Antitrust vengono descritte talune condotte tenute dalla SIAE ed in particolare l'esercizio di pressioni di vario genere per dissuadere gli autori a conferire mandato, anche solo per taluni diritti o servizi, ad altre *collecting*. Sembrerebbe inoltre che la SIAE starebbe minacciando e diffidando gli utilizzatori dal pagare a *collecting* diverse la quota parte di *royalty* loro spettanti, così da raccogliere anche i compensi spettanti ad autori o editori che non sono iscritti iscritti alla società, ed applicherebbe loro condizioni, economiche e non, diverse e più convenienti, determinando così ingiustificati vantaggi in favore di talune categorie di imprese, al fine di mantenerne in esclusiva i rispettivi compensi. Dalla documentazione prodotta emerge che la SIAE eseguirebbe di prassi richieste di *fee* di iscrizione anche ad autori non iscritti ad alcuna *collecting* o non iscritti alla SIAE bensì ad altre *collecting*, oltre a frapporre enormi ostacoli alla risoluzione del mandato dell'autore, anche solo per alcune opere o alcuni diritti o categorie di diritti, così da disincentivarne il passaggio ad altre *collecting*. Le chiedo, pertanto, di fornire a me ed ai colleghi cofirmatari un riscontro alle richieste sopra descritte ed alle altre riportate nei molteplici atti di sindacato ispettivo.

in materia di diritto d'autore, che è stata abbinata - come lei ha sottolineato - a interpellanze e interrogazioni analoghe presentate dalla senatrice Fucksia e dal senatore Crimi.

con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva n. 26 del 2014, prima richiamata, cosiddetta direttiva Barnier. Preliminarmente occorre ricordare che la suddetta direttiva - recepita in Italia sulla scorta degli specifici criteri di delega fissati dalla legge n. 170 del 2016, all'articolo 20 - ha introdotto principi utili a operare la più completa armonizzazione di *governance* delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore in Europa e a favorire la diffusione della musica *online* attraverso la concessione di licenze multi territoriali. Essa ha sancito, tra gli altri, il diritto del titolare dei diritti di autorizzare un organismo di gestione collettiva di sua scelta a gestire i diritti o le categorie di diritti per i territori di sua scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento dell'organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti; disposizione recepita all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35, in cui peraltro il legislatore italiano ha ricompreso anche le entità di gestione indipendente. Occorre ancora considerare che la particolare conformazione dei diritti di autore e connessi, le peculiari caratteristiche dei servizi erogati dagli intermediari, connotati da elevati costi fissi e da contenuti costi variabili, oltre alla varietà delle forme espressive della creatività, hanno favorito in tutta Europa la costituzione di situazioni di monopolio legale, naturale o di fatto. Che tali modelli economici siano tutti ugualmente legittimi e potenzialmente efficienti è un dato riscontrabile nella giurisprudenza europea e confermato dalla stessa direttiva 2014/26/UE, che non ha limitato gli Stati membri con riguardo all'attuazione dei modelli economici di gestione dei diritti. Inoltre, pur qualificando l'attività di intermediazione come fornitura di un servizio, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che l'articolo 16 della direttiva 2006/123/UE sulla libera prestazione di servizi non è applicabile alla materia dei diritti d'autore e connessi, per espressa esclusione operata dall'articolo 17 della stessa direttiva; ne consegue che la direttiva in parola, non essendo applicabile a questo tipo di servizi, non impedisce a una normativa interna di attribuire il monopolio legale del servizio a un ente. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, il legislatore italiano ha, in un primo momento, ritenuto prudente conservare una riserva legale in favore della SIAE per quanto riguarda l'attività di intermediazione dei diritti di autore, peraltro espressamente prevista dal legislatore in sede di emanazione dei principi di delega, e la totale liberalizzazione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha posto fine al monopolio del Nuovo IMAIE. In questo ultimo ambito - come è noto - a dimostrazione delle difficoltà incontrate, si è potuto registrare che la polverizzazione dei repertori e delle *collecting*, nonostante la regolazione amministrativa di dettaglio volta a disciplinare e riordinare la materia, ha determinato l'insorgenza di persistenti criticità, tra l'altro adesso richiamate dall'interrogante, che - si auspica - potranno trovare una risoluzione in forza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 35 del 2017 e dell'adeguamento delle *collecting* dei diritti connessi ai principi di trasparenza e di *governance* richiesti dalla normativa vigente. In tal senso strategico appare il ruolo di vigilanza attribuito dall'articolo 40 del decreto n. 35 all'Autorità di garanzia nelle comunicazioni. Con riferimento ai presunti profili di possibile incompatibilità di alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 35 con la direttiva 26 - come già espresso in altre recenti sedi e, in particolare, nella comunicazione effettuata il 12 settembre scorso da parte del ministro Franceschini e del sottosegretario per le politiche europee Gozi alla Commissione europea a seguito dell'incontro svolto a Venezia il 4 settembre, nella consueta ottica di collaborazione con la Commissione europea che sempre ha contraddistinto il Governo italiano, è stata espressa - penso che questo sia importante - la volontà di presentare in Parlamento un imminente intervento legislativo puntuale, che possa migliorare ulteriormente l'efficienza del sistema di gestione del diritto d'autore, al contempo raccogliendo certamente le istanze manifestate anche nelle interrogazioni riscontrate in questa sede - sono importanti come stimolo al Governo, che ha contezza della problema e voglia di trovare una soluzione condivisa - e volte a una liberalizzazione del settore della gestione collettiva dei diritti di autore. In tale prospettiva, coerentemente con l'impianto generale e con l'articolo 5 della direttiva in parola, il Governo intende proporre al Parlamento una disposizione che consenta in Italia, a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti nel territorio dell'Unione europea, non aventi fini di lucro e costituiti su base associativa, di poter procedere direttamente alla raccolta dei diritti, oltre che alla rappresentazione dei propri associati, eliminando la riserva di legge in favore della SIAE ed effettuando gli opportuni correttivi alla normativa vigente che assicurino una effettiva concorrenza. Relativamente alle denunciate inefficienze dell'ente, occorre innanzitutto evidenziare le nuove misure previste anche nel decreto legislativo n. 35, che definiscono una serie di stringenti criteri, una più serrata tempistica e forme di controllo più penetranti sulle attività di ripartizione, di riscossione, sull'impiego dei proventi e sui servizi offerti dagli organismi, nonché sulle modalità di distribuzione degli importi dovuti, al fine primario di garantire la piena trasparenza. Si deve, inoltre, rilevare che a partire dal rendiconto di gestione del 2011 tutti gli esercizi della SIAE si sono chiusi in positivo e anche l'ultimo rendiconto di gestione approvato dalle amministrazioni vigilanti ha registrato un avanzo di 984.913 euro rispetto all'anno precedente. non è sufficiente, ma è un dato da tenere in considerazione insieme ad altri. L'ente attualmente, ma anche e a maggior ragione alla luce delle svolte normative e competitive annunciate, è comunque già stato chiamato a conformarsi agli *standard* di *governance*, di efficienza e trasparenza previsti dalla direttiva e volti a garantire la migliore tutela dei titolari dei diritti. Con riferimento alle richieste di istituire una Commissione ministeriale ovvero un tavolo tecnico, allo scopo di monitorare lo stato della SIAE, stanti le considerazioni sopra svolte sulle evoluzioni intervenute, in particolare in materia di trasparenza e controlli, atteso che l'ente è sottoposto, per effetto della legge n. 2 del 2008, alla vigilanza permanente e congiunta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di specifica competenza, a cui si aggiungono, a far data dall'11 ottobre prossimo venturo, le funzioni di vigilanza e ispettive affidate all'Agcom sul rispetto delle disposizioni normative (articolo 40 del decreto legislativo n. 35 del 2017), sembra opportuna una preliminare verifica delle ulteriori attività di controllo già in corso di implementazione. In conclusione, in risposta ai senatori interroganti e interpellanti, si ritiene che il Governo abbia negli ultimi anni intrapreso importanti iniziative per una gestione efficiente e trasparente dei diritti d'autore e dei diritti connessi. Si intende proseguire in questo senso, anche con l'intervento di ulteriore liberalizzazione preannunciato, proseguendo nel confronto con le istituzioni europee e con il Parlamento nazionale - in quest'ottica ben vengano sollecitazioni come quella di oggi pomeriggio per disciplinare al meglio un settore tanto importante per la crescita economica e culturale del Paese, in considerazione della primaria esigenza di garantire pienamente la tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.

come ricordato dalla collega Fucksia - quando parlavano per noi De Amicis o Giuseppe Verdi. Ovviamente il mondo è cambiato molto da quel momento e certamente, lei non trova di fronte una persona che vede la liberalizzazione in sé come taumaturgica risolutrice di tutti i mali. Anzi, vorrei dire che, quando parliamo di previdenza e di diritti, dobbiamo prestare la massima attenzione. Ma l'interlocuzione che c'è stata con il Governo nel corso degli ultimi mesi ha portato all'evidenza il fatto che dobbiamo saper coniugare la necessità di garantire - così come prevede la disposizione europea

così antiquato e vetusto per l'aspetto relativo del vincolo, andando ad esentare progressivamente dall'obbligo del bollino SIAE, un retaggio in qualche modo anacronistico, anche per le modalità con il quale viene ancora applicato.

che premono e che obiettivamente hanno la loro ragione per farlo, affinché effettivamente gli autori, gli scrittori, i cantanti e i musicisti italiani possano scegliere la migliore gestione possibile in relazione anche alle loro necessità future.

chiedo di accelerare per quanto possibile la piena armonizzazione del nostro diritto rispetto al tema dei diritti degli autori

CRIMI *(M5S)*. Signor Sottosegretario, mi passi la battuta: ascoltando la sua risposta si può dire che per la SIAE la musica rimane sempre la stessa.

rimarcare il fatto che esiste una distinzione netta tra gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente. È lì che nasce tutto. Dal decreto legislativo n. 35 del 2017, da lei citato, nel recepire la direttiva europea, ha introdotto ha introdotto la seguente precisazione: mentre la direttiva europea semplicemente dice che ogni titolare di diritto può rivolgersi a un qualunque organismo di gestione collettiva, voi avete tenuto a precisare «o a un'entità di gestione indipendente», distinguendo i due casi e facendo alla fine salvo quanto già disposto dalle leggi precedenti in merito al monopolio SIAE. Quello che probabilmente si delinea dalle parole che

di collaborazione già consolidati nel tempo. Si tratta, quindi, di una falsa liberalizzazione. L'opportunità verrà invece negata agli operatori organizzati diversamente dalla SIAE, quelli che rappresentano gli artisti sulla base di mandati commerciali e, quindi, in forma non collettiva,

della SIAE. Gli artisti e gli utilizzatori che nei mesi scorsi hanno lasciato la SIAE - siamo a circa 8.000 - per le alternative da loro considerate più idonee, continueranno così a operare in una situazione di incertezza giuridica pressoché totale. Quindi, avremo, da una parte, la SIAE che intima di non pagare

un fatto. Tutti gli sforzi per mantenere il monopolio SIAE sono inutili: ormai le stalle sono state aperte e i buoi sono scappati. Gli autori hanno abbandonato la SIAE e sono già 8.000 coloro che si sono iscritti presso altri soggetti, tra cui personaggi di un certo rilievo.

Se leggiamo le ordinanze di ripartizione di compensi a favore di autori ed editori, non troviamo traccia chiara dei meccanismi di ripartizione di quei proventi. Ci chiediamo se quei profitti e quel valore vengono redistribuiti con gli autori ed editori, e parliamo di un flusso di soldi molto importante (forse quello che genera oggi gli utili della SIAE). Quando discuteremo la legge di stabilità, il Movimento 5 Stelle sarà lì a porre la lente di ingrandimento su questo tema insieme all'ampio arco parlamentare qui rappresentato. Gli artisti sanno che ci sono alternative e devono avere il diritto di scegliere.

A oggi gli organismi di gestione collettiva hanno sottoscritto già degli accordi di rappresentanza in virtù dei quali SIAE raccoglie in Italia i compensi degli artisti stranieri, mentre all'estero le *collecting* come la SIAE raccolgono per gli italiani. Quindi, le previsioni

La modifica normativa, prevista anche in previsione della legge di bilancio, appare sinceramente una beffa, che segue il grave danno arrecato sia ai titolari dei diritti, sia agli utilizzatori. Il tema vero è invece redigere criteri oggettivi per stipulare accordi di rappresentanza equi e non discriminatori, anche per le entità di gestione indipendente e, comunque, nelle more, consentire che la raccolta dei compensi possa essere svolta non solo dai singoli autori, ma anche dagli aventi causa di questi, ivi esclusi gli enti di gestione indipendente. Pertanto, la soluzione appare tutta in divenire e si spera che, con delle disposizioni di legge precise, si vada a sanare la situazione, in